Signor Presidente, onorevoli senatori, con questa interrogazione

Ricordo che la manifestazione nazionale era stata indetta dal Consiglio nazionale dei geologi ed aveva come fine quello di promuovere la "riforma delle libere professioni, contro il c.d. decreto Bersani". Al previsto corteo, snodatosi da piazza del Colosseo a piazza Madonna di Loreto, a cui hanno partecipato, tra gli altri, numerosi parlamentari, prendevano parte oltre 10.000 persone, appartenenti a varie categorie di liberi professionisti, quali geologi, architetti, ingegneri, avvocati, commercialisti, medici, farmacisti e così via. In piazza Madonna di Loreto, ove era stato installato un palco per gli interventi, erano stati altresì predisposti adeguati sbarramenti, presidiati dalle forze di polizia, per evitare che - come successo in passato - i manifestanti, eludendo i controlli, si dirigessero alla spicciolata verso Palazzo Chigi. Era stato peraltro consentito, nel contempo, il transito ai mezzi di soccorso ed ai parlamentari di rientro dall'evento. Momenti di tensione si sono verificati allorquando il personale delle forze dell'ordine ha evitato, come peraltro avvenuto in occasione di precedenti manifestazioni svoltesi anche durante la passata legislatura, che la pressione esercitata dal corteo consentisse ai partecipanti di giungere a Palazzo Chigi, dove in quel momento era in corso il Consiglio dei ministri. Al termine degli interventi, alle ore 13,30 circa, vi è stato un rapido deflusso dei manifestanti verso via dei Fori Imperiali e via Nazionale. Preciso che, pur essendosi impedito con fermezza ad alcuni gruppi di partecipanti alla manifestazione di procedere in direzione di via del Corso, non vi è stato alcun episodio di violenza e non è mai stato interrotto il traffico veicolare in piazza Venezia, nel tratto che va da via Nazionale che va da via Nazionale al Teatro di Marcello, ed è sempre stato consentito - come è giusto - il libero movimento dei parlamentari. Ribadisco, inoltre, che anche nel corso di questa manifestazione sono stati adottati i criteri di ordine pubblico previsti per tutte le manifestazioni che si svolgono nella capitale e che interessano il centro storico. Ricordo, infine, che, anche nelle situazioni più delicate, il Ministero dell'interno e le forze dell'ordine hanno come fine prioritario quello di garantire la libertà di manifestazione, salvaguardando, nello stesso tempo, l'ordine pubblico ed anche la sicurezza di tutti i cittadini, manifestanti e non. Credo di poter dire che questo compito difficile, che richiede grande professionalità, è stato assolto in maniera corretta e rispettosa dei diritti fondamentali prescritti dalla Carta costituzionale.

vorrei semplicemente far rilevare al rappresentante del Governo, che ringrazio e a cui rivolgo anche un augurio e un saluto

essere stato predisposto per impedire ai manifestanti di recarsi a Palazzo Chigi, abbiamo chiesto ai

perché, signor Vice ministro, la comunità è sconcertata da alcuni atteggiamenti assunti dal Governo. Ci troviamo in presenza di una finanziaria che sta riscuotendo dissensi da tutte le parti; è un provvedimento che non ha accontentato nemmeno una categoria produttiva. Domenica scorsa, sono stato invitato ad un'assemblea

Quindi, dobbiamo immaginare che, anche in futuro, altre categorie produttive potranno scendere in piazza, come è giusto fare, in maniera pacifica e non violenta, per far sentire la propria voce.

denotanti la caratteristica di un'opera ad alto valore reddituale, capace di autofinanziarsi come attestato da grandi *advisors*.

che ha individuato il *general* *contractor.* Mi sembra quindi veramente autolesionista per un Paese che immagina uno sviluppo armonico del suo territorio e vuol consentire a tutte le sue comunità eguali possibilità di sviluppo, mettere in discussione e compromettere questo progetto in modo definivo. ha un bel dire il Governo quando definisce la non priorità di quest'opera, non avendo giustamente il coraggio di affermarne il disvalore, perché metterebbe in imbarazzo il Presidente del Consiglio dei ministri,

post-ideologiche o forse ancora ideologiche dei Ministri dei trasporti e dell'ambiente per definirla come l'opera più dissennata mai pensata in questo Paese, il più grande spreco di risorse, la più inutile e dannosa opera mai progettata in Italia.

nella sua individuazione originaria, nel suo *excursus* procedimentale e perfino nella definizione degli atti contrattuali. Davvero un Paese impazzito, se oggi bastano le espressioni così determinate ed

di qualche Ministro? Mi pare che su questa grande infrastruttura sia stata compiuta un'opera di mistificazione ideologica. Si è costruito, ad esempio, un meccanismo di comunicazione che l'ha descritta come un'opera inutile quando invece è un'opera essenziale per la possibilità di attivare veramente una connessione infrastrutturale importante, che può consentire di realizzare una piattaforma logistica integrata nell'area siculo-calabrese, consegnando a quei territori e a quelle comunità

sviluppando, utilizzare al meglio gli approdi siciliani, le grandi potenzialità di un'industria agroalimentare in grande sviluppo e anche la grande vocazione turistica di quel territorio, con l'effetto volano

positivo sul piano del suo valore strategico da misurarsi con il mercato e da pretendere di utilizzare le regole di mercato per il suo finanziamento.

prevalente del finanziamento era stato rintracciato sul mercato dei capitali attraverso due *ad**visor* che stavano operando in tal senso. Quindi, un'opera per larga parte

economica, in termini di sviluppo, che contraddice questa opera. Vi è soltanto una presa di posizione ideologico-politica; ci pare un prezzo troppo che le popolazioni siciliane e calabresi devono pagare. Vorrei che fosse il Governo, con un atto di umiltà, a rivolgersi a quelle popolazioni. Come vuol fare per l'area del Nord-Ovest, per la Val di Susa, legittimamente, chiedendo il conforto di quelle popolazioni o, comunque, assistendole con una serie di rassicurazioni importanti che possono consentire di realizzare quella grande opera strategica in termini di sicurezza e di ecocompatibilità. Anche su questo terreno il Ponte sullo Stretto è stato immaginato con tutte le garanzie e le tutele di ecocompatibilità. Volete poi considerare anche il valore simbolico, la sfida tecnologica di una grande opera che venisse ad insediarsi nella area più marginale di questo Paese? Quale valore d'impatto ha un'opera come quella rispetto alla alla percezione che si ha del sottosviluppo, dell'arretratezza di quei territori e di quelle popolazioni? Una grande sfida tecnologica, la più alta al mondo che si compie nella terra che forse rappresenta in modo più emblematico la contraddizione di questo Paese e del suo sottosviluppo, che non può essere accettata in modo perenne dalle nostre popolazioni. È una vicenda che la politica dovrebbe misurare in termini diversi, sottraendola al confronto ed allo scontro polemico e consegnandola ad un confronto più civile, più sereno, chiamando in causa anche le popolazioni. Vedete, abbiamo confidato che vi fosse un ascolto maggiore. Abbiamo organizzato manifestazioni popolari; ne abbiamo già fatte per rendere evidente quanto elevato sia l'interesse rispetto a quest'opera.

chiudere questa partita, altro che non prioritaria! Interrompere la procedura relativa ad una gara già espletata significa per anni questa grande opera: una grande opera come il Ponte sullo Stretto non può essere riattivata in termini brevi. Se viene interrotta nel suo percorso, verrà consegnata agli archivi, alle scartoffie, verranno sprecate risorse e probabilmente sarà pagata anche una costosissima penale; sarà impedita un'iniezione di sviluppo. Anche l'operazione di ripartire le risorse ai territori mi sembra davvero ridicola (scusate il termine un po' irrituale), perché un'opera di questo impatto, quanto meno di 6 miliardi di euro, viene cassata, ma il miliardo è più di euro di FI\NTECNA viene ripartito, secondo criteri geopolitici tra le due aree interessate, attraverso un meccanismo particolarmente complicato, con un decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con quello dell'ambiente e dell'economia, sentite le Regioni interessate.

che il Mezzogiorno ha bisogno di ben altri investimenti per ridurre il divario infrastrutturale drammatico, che anche l'ultima legge-obiettivo ha ulteriormente aggravato con una ripartizione delle risorse finanziarie assolutamente sproporzionata tra le aree del Nord quelle del Centro, del Mezzogiorno e della Sicilia in modo particolare. Sappiamo di venire da una condizione di grande debolezza, ma ad una debolezza non si reagisce addirittura aggravandola ulteriormente. Avremmo preteso il rispetto di una procedura contrattuale assolutamente legittima e ulteriori investimenti in infrastrutture che potessero consentire a questi nostri territori di avere le medesime opportunità di sviluppo.

un sistema di Governo di questo Paese, trattandosi di investimenti dello Stato nazionale, dello Stato centrale, di grandi enti economici? Guardate il livello di investimenti che l'ANAS o Ferrovie dello Stato Spa hanno destinato al Mezzogiorno o al Centro-Nord;

Non vedo le ferrovie; non vedo l'alta velocità; non vedo l'alta capacità né l'intermodalità; non vedo neanche i finanziamenti per il completamento dell'anello autostradale siciliano. Non vedo il raddoppio della Catania-Ragusa, né quello della Catania-Gela, la strada della morte,

abbiamo un'altra possibilità. Ho presentato anche una mozione al Senato nella quale torno a dire le stesse cose. Spero che l'equilibrio così risicato del Senato

Forse quest'opera, sottratta agli schieramenti, potrebbe diventare la grande occasione per un territorio che ha bisogno di una grande prospettiva di crescita e di sviluppo.

alla Camera dei deputati varie risoluzioni che hanno determinato un dibattito politico e alla fine anche un voto.

di ordine ideologico, non è che ci sono due ministri che hanno imposto che il ponte non s'ha da fare. Vorrei solo ricordare che la questione del ponte era inserita nel programma Prodi durante la campagna elettorale: si tratta quindi di una posizione assunta antecedentemente sia al risultato elettorale che alla costituzione del Governo. costituzione del Governo. La differenza è, secondo me, di ordine anche filosofico. C'è una filosofia. C'è chi ritiene che una grande opera o una grande infrastruttura bisogna collocarla a prescindere dal contesto;

Ecco perché consideriamo il ponte sullo Stretto un'opera non inutile, ma non prioritaria rispetto ad altri progetti che pensiamo

e nei confronti di due Regioni quali la Calabria e la Sicilia. Qual è l'attenzione che il Governo pensa di mettere in campo per queste due Regioni?

ponte? Il problema è che il ponte viene più immaginato come un'opera che attrae turismo piuttosto che come un mezzo per collegare i due continenti. Non è vero che noi

Se immagino per la Sicilia, la Calabria e il Mezzogiorno d'Italia il medesimo *trend* di crescita di questi anni, di questi decenni, di questo secolo e mezzo di unità d'Italia, so che il divario non sarà mai colmato e che questo sarà un Paese spaccato a metà in modo irreversibile,

Se questo Governo, quello precedente, quello ancora prima, crede davvero che una vocazione di questo nostro Paese sia quella del partenariato euromediterraneo (che dal 1992 ad oggi non è mai stato assistito da alcuna politica di vera cooperazione allo sviluppo), di avere rapporti con quest'area, che è il vero bacino di riferimento in cui il nostro Paese può essere un *leader*, ebbene, io ho guardato con grande apprezzamento alla scelta di misurarci

Il vero destino di questo nostro Paese è di riprendersi un ruolo di centralità e di *leadership* nel Mediterraneo, quindi è opportuno infrastrutturare il Mezzogiorno. In questo modo, se immaginiamo la Sicilia come punto più avanzato, che intercetta le merci e i grandi flussi che arrivano dal Sud-Est asiatico e da un Nord Africa che si svilupperà, il Ponte serve.

2.500 anni di storia, che vanno dalle vestigia della Magna Grecia alle opere della modernità, che registra un flusso turistico in grande crescita, il Ponte costituisce di per sé un valore

perché, essendo un progetto che è stato approvato dall'Unione Europea nell'ambito della *start list*, è oggetto di cofinanziamento fino al 20 per cento. Il precedente Governo aveva contrattato e definito questa intesa, inserendo nella *start list* il ponte sullo Stretto. Con una scelta diversa, immagino che il Paese

Con la legge n. 93 del 2001 il Parlamento decise di istituire il Parco nazionale della Costa teatina che insiste su un tratto di costa abruzzese, in particolare della Provincia di Chieti, ben conservato e di grande pregio ambientale e naturalistico. La Regione ebbe ad impugnare la legge avanti la Corte costituzionale, ritenendo essere stata invasa la sua potestà legislativa quanto ai profili di tutela del territorio, ma la Corte costituzionale, con pronuncia del 2002, rigettò l'istanza ritenendo la questione sollevata dalla Regione Abruzzo non fondata, così che la legge continuò ad avere vigore. A distanza di oltre cinque anni e mezzo dall'approvazione della legge di cui sopra e di circa quattro anni dalla pronuncia della Corte costituzionale, questo Parco ed alcuni altri previsti dalla medesima disposizione di legge non risultano istituiti. La ragione sembra chiara agli interpellanti e a chi parla e naturalmente è da ricondurre alle opzioni politiche e all'indirizzo programmatico sia del passato governo regionale abruzzese, di centro‑destra fino al 2005, che ebbe

di istituire ‑ come è noto ‑ nuove aree protette di rilevanza nazionale, tra cui il Parco della «Costa teatina». Stante il mutamento d'indirizzo politico sia a livello regionale che nazionale e stante la vigenza della legge in questione, che autorizza l'istituzione del Parco, si trattava e si tratta - è questo il senso dell'iniziativa - di accertare in modo chiaro con un atto di sindacato ispettivo nell'Aula parlamentare del Senato della Repubblica la volontà del Governo

tra il Ministero e la Regione, ma riteniamo utile questo atto parlamentare finalizzato - ripeto - ad acclarare la volontà del Governo nel senso auspicato. L'istituzione del Parco, che, per la verità, fino a qualche tempo fa non era diffusamente sostenuta dagli enti locali e dal territorio, oggi invece è molto rivendicata dai sindaci e dalla popolazione, anche perché da alcuni mesi è stato dismesso il vecchio tracciato ferroviario che segue il tratto di costa in questione e le aree di risulta, che si presentano estese e di grande pregio e valore, valore, sono oggetto di attenzione da parte di privati ma anche, per fortuna, da parte degli enti locali, della Provincia di Chieti e dei Comuni interessati (circa dieci), che si sono candidati a rilevare la proprietà dei siti coinvolti, anche per evitare tentativi speculativi, con una procedura che si sta svolgendo di concerto con RFI e che attualmente è in fase di definizione. L'istituzione del Parco nazionale in commento aiuterebbe anche a pianificare e programmare l'uso di tali preziose aree di risulta. Si tratta, altresì, di verificare la sostenibilità finanziaria dell'istituzione del Parco nazionale della Costa teatina, anche alla luce delle notevoli decurtazioni di fondi destinati alle aree protette che si è verificata negli esercizi finanziari pregressi. È quindi evidente che la volontà che eventualmente il Governo, per mezzo del sottosegretario Dettori oggi presente in Aula, volesse esprimere andrà accompagnata anche da uno sforzo finanziario, per la verità di dimensioni non

sfuggito alla speculazione edilizia che ha caratterizzato invece diversi altri estesi tratti di costa abruzzese, e non solo abruzzese. Esso presenta caratteristiche ambientali di grande rilevanza, come la presenza di oasi e di emergenze naturalistiche talvolta eccezionali. È uno dei tratti di costa più belli dell'Adriatico e merita uno strumento di tutela e sviluppo che solo l'istituzione di un parco di rilevanza nazionale gli può attribuire. Come dicevo prima, so che la Regione non ha ancora formalizzato una proposta di perimetrazione, ma spero e credo che ciò potrà essere fatto nel caso in cui il Governo, come mi auguro, voglia oggi qui esprimere un chiaro e netto orientamento nel senso

mi corre l'obbligo lasciare agli atti la cronistoria di questa vicenda, per cui adempirò il mio compito

In merito a quanto rappresentato con l'interpellanza 2-00041, dal senatore Legnini ed altri senatori, relativa all'istituzione del Parco nazionale della Costa teatina, si rappresenta che la procedura per l'istituzione del parco in oggetto era stata avviata, come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 8 marzo 2001, n. 93. La Regione Abruzzo ha adito la Corte costituzionale, in data 3 maggio 2002, per richiedere una dichiarazione di illegittimità costituzionale di tale norma, in quanto ritenuta lesiva delle prerogative e delle attribuzioni della Regione stessa. In pendenza di tale ricorso e in attesa di un suo esito, l'attivazione del procedimento istituivo del Parco era stata quindi sospesa. In seguito alla dichiarazione di non fondatezza della questione di incostituzionalità della norma da parte della Suprema corte, intervenuta con sentenza n. 422 del 7 ottobre 2002, la direzione per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente ha convocato una riunione, in data 16 gennaio 2003, al fine di avviare il procedimento amministrativo di istituzione del Parco nazionale in oggetto. I rappresentanti della Regione e della Provincia che hanno partecipato alla predetta riunione hanno espresso il mandato, ricevuto dai rispettivi presidenti, di ritenere l'istituzione del Parco in esame incompatibile con quanto previsto nel documento quadro di riferimento regionale, deliberato dal Consiglio regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale regionale il 24 marzo 2000. Si sono dichiarati disponibili ad avviare una concertazione solo nell'ipotesi di lavorare ad un progetto speciale territoriale, così come previsto nel documento citato, e si sono dichiarati non favorevoli ad avviare il procedimento di istituzione di un ente Parco nazionale. In data 4 aprile 2003 la direzione per la protezione della natura ha inviato al Ministro dell'ambiente *pro* *tempore* una nota, nella quale era stata avanzata la possibilità di sensibilizzare la Regione a collaborare per l'istituzione del Parco, sottoponendogli alla firma una nota in tal senso, in considerazione del fatto che l'istituzione di un ente Parco nazionale, secondo lo schema normativo, non può prescindere dall'intesa con la Regione territorialmente interessata. Ogni attività tendente alla realizzazione del Parco cessava in tale data. Un nuovo interesse al Parco è stato rappresentato dalla Regione Abruzzo con la nuova amministrazione regionale insediatasi nel 2005. L'interesse, però, non è stato mai riscontrato con gli enti locali sulla base di una perimetrazione possibile. Ciò nonostante, in considerazione del fatto che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha ancora particolare interesse affinché il Parco venga istituito, in data 6 settembre 2006 si è svolta nella sede ministeriale un incontro con i rappresentanti della Regione Abruzzo ed in particolare con l'assessore all'ambiente di questa. Nel corso della riunione è stato raggiunto un accordo in base al quale la Regione Abruzzo, al fine dell'avvio del procedimento di istituzione del Parco nazionale, sottoporrà all'amministrazione che rappresento una prima ipotesi di perimetrazione dell'area protetta. Ad oggi, questa ipotesi di perimetrazione non è ancora pervenuta. A conforto di quanto gli interroganti mettono a disposizione, voglio aggiungere che l'attenzione sull'istituzione di nuovi parchi e nuove aree protette da parte del Governo e del Ministero che rappresento è molto alta. Certo, si tratta di istituire queste zone con la denominazione «parco» non contro i territori, ovviamente, né contro chi abita questi territori. La sensibilità che abbiamo riscontrato in questo ultimo approccio al problema è molto alta e in questa direzione ci stiamo muovendo. Quella della tutela ambientale è una scelta strategica, a cui tutti stanno guardando con grande interesse, perché rappresenta il vero futuro del nostro Paese. Corrispondere alle istanze dei territori senza prevaricarne pertanto gli atteggiamenti e le scelte è compito assai delicato. Questo Governo credo di interpretarne in tutta la sua dimensione questo aspetto - intende sviluppare ogni iniziativa per favorire la nascita di questi parchi, non parchi, non solo in termini procedurali, ma anche in termini sostanziali, mettendo anche a disposizione risorse. Senza queste ultime, infatti, è chiaro che i territori si trovano svantaggiati nell'impostazione complessiva del problema. Per quanto mi riguarda - ma

Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario, professor Dettori. Dichiaro di essere molto soddisfatto della risposta del Governo all'interpellanza sottoscritta da chi parla e da altri 36 colleghi senatori. La risposta dimostra La risposta dimostra una chiara volontà politica del Governo, e per esso del Ministero dell'ambiente, di provvedere all'istituzione del Parco nazionale della «Costa teatina». Abbiamo potuto accertare, con la risposta testé ascoltata, che fino ad oggi, come si paventava nell'atto di interpellanza, il Parco non è stato istituito per difetto di concerto tra la Regione Abruzzo e il Ministero stesso. Tale Regione è stata governata dal centro-destra fino al 2005; è quindi chiara la ragione per la quale ad oggi questa volontà legislativa non risulta attuata. non risulta attuata. Come dicevo nel precedente intervento, ora potrà attivarsi questa procedura di concerto tra la Regione e il che, come diceva il Sottosegretario, è assolutamente necessaria per definire la procedura e per provvedere alla concreta istituzione dell'ente Parco, coinvolgendo gli enti coinvolgendo gli enti locali. Sono particolarmente d'accordo con la sottolineatura che faceva il Sottosegretario a conclusione della sua risposta, laddove egli egli evidenziava l'assoluta necessità di coinvolgere gli enti e le popolazioni locali non soltanto nella fase istitutiva, quindi nella fase di perimetrazione (che peraltro non è semplice, trattandosi di un territorio urbanizzato e di una costa sulla quale insistono diversi centri urbani), ma anche nella fase di vita e di gestione di questo Parco, come di tutti i parchi nazionali. Mi conforta, infine, l'affermazione in base alla quale è intenzione del Governo riprendere e ridare vigore a una politica seria sulle aree protette, munendole delle risorse finanziarie che in questi anni sono mancate e che hanno determinato un'asfissia gestionale degli enti medesimi, svuotandone le potenzialità non soltanto relativamente alle esigenze di tutela e di protezione della natura, ma anche per quel che riguarda il loro ruolo, finalizzato a dare impulso allo sviluppo dei territori interessati. Credo, quindi, che l'atto che abbiamo presentato e, soprattutto, la risposta del Governo, possano mettere un punto fermo nell'acclaramento della volontà del Governo stesso e possano consentire di